dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonche´ ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Prima di iniziare i lavori di questo pomeriggio, ritengo doveroso rivolgere il nostro pensiero alla tragedia che la notte scorsa si everificata lungo l’autostrada A16, in provincia di Avellino. In questo momento di lutto e di sofferenza, desidero innanzitutto far giungere ai familiari delle 38 vittime l’accorato cordoglio di tutti noi, unitamente agli auguri di pronta guarigione per i dieci feriti coinvolti in questa terribile sciagura. Lo sgomento per quanto verificatosi non deve trattenerci dal fare chiarezza sull’accaduto. E[ ]necessario che le autoritacompetenti utilizzino tutti i poteri a loro disposizione per accertare le cause dell’incidente, perche´ vengano verificate le eventuali responsabilita e perche´ simili eventi non abbiano piua ripetersi. In Italia gli incidenti stradali continuano a rappresentare una tra le principali cause di morte. Abbiamo il dovere morale di intervenire intensificando i controlli sui conducenti dei veicoli ed in particolare su coloro che svolgono quest’attivita a titolo professionale, monitorando con estremo rigore le condizioni di sicurezza dei veicoli, la qualita` tecnica dei tracciati stradali, delle barriere di protezione.

come ormai tutti sanno, una tragedia di immani proporzioni in termini di vite umane eaccaduta intorno alle 20,30 di ieri, quando un pullman con 50 persone a bordo e precipitato da un viadotto

Il bilancio ufficiale parla di 39 vittime estratte dai vigili del fuoco – ai quali va il nostro piu vivo ringraziamento per quello che hanno fatto, insieme alle forze dell’ordine, come detto prima dal presidente Grasso – che hanno estratto dalle lamiere dell’autobus undici superstiti, tutti purtroppo feriti. Non eil Non eil primo incidente che si verifica in quel tratto autostradale, ritenuto da sempre pericolosissimo. Tutti, rappresentanti delle istituzioni, cittadini della provincia di Avellino, della regione Campania Campania e dell’Italia intera, ci sentiamo profondamente colpiti da quanto e accaduto e ci sentiamo vicini ai familiari e agli amici delle vittime. Mi risulta che proprio in queste ore rappresentanti del Governo si stanno recando presso la scuola media di Monteforte Irpino, dove, dalla notte di ieri, estata allestita una camera ardente. A tutti i A tutti i familiari va la piu sentita vicinanza, mia personale, di tutto il Gruppo parlamentare del Popolo della Libertae dei parlamentari del Popolo della Liberta della regione Campania. (Applausi Presidente, vorrei associarmi al profondo cordoglio e e dolore che ha colpito tutta l’Italia e, in particolar modo, la Campania. Sono vicino anche all’ex presidente della Provincia Sibilia, con il quale ci conosciamo benissimo, essendo entrambi campani.

Giugliano in Campania e da Marano di Napoli, zone vicinissime a noi. Credo che noi del Senato dobbiamo far sentire la nostra vicinanza alle famiglie.

che portano a Pietrelcina, ci sono tantissimi agriturismi e molte persone in questo periodo preferiscono il fresco di un agriturismo alla calura del mare. Quindi, occorre stare attenti

esprimiamo vicinanza anche nei confronti dei Vigili del fuoco e delle Forze dell’ordine che in questo momento stanno facendo di tutto

che percorrono le nostre strade sono inadeguati: molto spesso non sono sicuri e soprattutto non sono controllati come dovrebbero

io sono di Pozzuoli e quasi tutte le vittime erano residenti nel comune di Pozzuoli e, quindi, come capirete, sento maggiormente questo triste evento.

accade sulle strade italiane, non semplicemente in tema di sicurezza, che pure e una questione centrale, ma anche riguardo alle condizioni di lavoro cui spesso sono sottoposti coloro che guidano autobus, camion, mezzi di lunga percorrenza.

sulla luciditadi chi guida un mezzo pesante. Naturalmente per noi questo e un tema di riflessione perche´ riguarda direttamente la capacita` del legislatore di intervenire anche su un tema come questo. La ringrazio e naturalmente mi associo al dolore delle famiglie.

Credo che quello che ci unisce sia il cordoglio, una riflessione sulle famiglie dilaniate, sui gruppi di amici che sono stati completamente disgregati in questo fatale incidente, irripetibile per quanto riguarda le dinamica, e che richiede da parte di tutti, sempre, un rigore, non eccessivo ma dovuto, per quanto riguarda la prevenzione. Mi Mi associo, signor Presidente, anche alle parole che ha voluto richiamare per quanto riguarda gli interventi delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco, dei volontari, dei medici e di quanti stanno cooperando

recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche´ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (890)

onorevoli colleghe e colleghi, signor Ministro, queste riflessioni sono a margine della discussione e si aggiungono a quelle che sono state esposte dai relatori nell’ultima seduta. Devo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti per i suggerimenti e per le critiche che sono state portate al provvedimento,

non si conclude con questo decreto-legge che, in larga misura, riguarda la lotta alla disoccupazione giovanile: altri interventi sono in programma,

Devo aggiungere poche parole a quelle gia espresse dai relatori per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge. Come i colleghi sanno, esso disciplina vari aspetti delle politiche del lavoro, e in particolare delle politiche attive: equesto il caso degli incentivi alle assunzioni di giovani con contratto a tempo indeterminato. Si vuole in questo modo favorire l’occupazione stabile

lo si faraquando saranno disponibili ulteriori risorse da dedicare alla riduzione del costo del lavoro, che rappresenta la variabile cruciale su cui intervenire per facilitare l’occupazione, soprattutto dei giovani. Il decreto-legge interviene anche sulle norme che regolano i contratti di lavoro: si tratta di materia complessa e delicata, su cui si manifestano i maggiori contrasti tra le forze politiche e le forze sociali. Nel corso della discussione alcuni senatori hanno criticato il decretolegge perche´ avrebbe aumentato eccessivamente la flessibilita; altri senatori lo hanno criticato per il motivo opposto, ovvero perche´ non avrebbe aumentato abbastanza la flessibilitanei rapporti di lavoro. ]vero che qualche forma di flessibilitae stata introdotta, ad esempio nei contratti di lavoro a tempo determinato, per lo piurinviando la materia alla contrattazione collettiva.

per quanto temporanei, offrono ai lavoratori e ai giovani le garanzie di legge e di contratto tipiche dei contratti a tempo indeterminato e che, in queste circostanze, potrebbero svolgere utilmente una funzione importante: quella di interrompere i lunghi periodi di disoccupazione e di inattivita, che sempre piuspesso colpiscono i giovani senza lavoro. D’altra parte, gli incentivi che vogliono

Il decreto-legge interviene poi su altre tipologie di contratti di lavoro temporaneo, come il lavoro intermittente e quello a progetto, per porre rimedio ad alcune carenze gia dimostrate dalla legge n. 92 del 2012.

Non si evoluto riaprire il confronto a tutto campo su questa materia e non si esclude di approfondirne in seguito ulteriori aspetti, tenendo conto del fatto che e tuttora in corso un’attivitadi monitoraggio sugli effetti della riforma, di cui si attendono i risultati. Si terra conto anche dei risultati di alcuni importanti negoziati che si stanno svolgendo tra le parti sociali a margine dell’attivitadell’Expo di Milano, che potrebbero portare a risultati importanti sui temi sia della flessibilita che della sicurezza dei lavoratori; risultati che possono dare utili indicazioni per essere, almeno in parte, ripresi ed estesi ad altri settori ed ambiti territoriali del Paese. Il Governo eimpegnato a seguire con attenzione queste vicende milanesi e a farne oggetto di confronto con le parti sociali a livello nazionale per individuare possibili evoluzioni e un rafforzamento delle norme incluse nel presente decreto. Ma forse la parte piu significativa del presente decreto, per lo meno per gli articoli che riguardano i temi del lavoro, consiste negli interventi a favore della cosiddetta occupabilitadei giovani, vale a dire la capacita dei giovani ad affrontare con maggiore probabilitadi successo la ricerca di un posto di lavoro stabile e qualificato. si osserva la costituzione di una struttura che il Governo vuole formare per affrontare il problema dei servizi per l’impiego, un problema affrontato dal Presidente del Consiglio in un question time tenuto al Senato Su questo terreno siamo molto arretrati: dobbiamo recuperare il terreno perduto velocemente; non sara facile, ma occorrerafare uno sforzo enorme, soprattutto se si vorra trarre vantaggio da quel programma per i giovani che la Commissione europea ci raccomanda e che vuole attuare a partire dal prossimo anno. Inoltre, il decreto contiene anche misure di contrasto alla poverta, soprattutto nel Mezzogiorno. Vanno altresı ricordate le norme in tema di start up e di facilitazione ulteriore per l’autoimprenditorialita`.

il decreto entra anche nella materia fiscale con il posticipo del pagamento dell’IMU e il rinvio dell’aumento dell’IVA. Sono risposte temporanee e parziali: verrail tempo per trovare soluzioni piu solide e condivise,

sistema tributario e contabile dello Stato, previdenza sociale e coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, riconducibili tutti alla competenza esclusiva dello Stato secondo, lettere e), o) e r) della Costituzione), nonche´ la materia tutela del lavoro, riconducibili alla potesta` legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni (articolo 117, terzo comma della Costituzione), esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che: a) sia soppresso il comma 17 dell’articolo 1, dal momento che la disposizione, nell’escludere che la decisione regionale in materia di incentivi possa prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quanto giaprevisto alla norma statale, e suscettibile di comprimere l’ambito di intervento riservato in materia alla competenza regionale; sia soppresso il comma 4 dell’articolo 2 in quanto la disposizione ivi prevista, incidendo in misura diretta sulla materia dei tirocini formativi, viola la competenza legislativa residuale delle Regioni, di cui all’articolo 117, quarto comma della Costituzione; c)

permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: sull’emendamento 01.2 parere non ostativo, nel presupposto che al comma 3 il coordinamento delle iniziative regionali e territoriali per l’occupazione, oggetto del piano pubblico definito dalla Conferenza nazionale per il lavoro, non incida sull’autonomia normativa e finanziaria di Regioni ed enti locali. Si segnala, inoltre, al comma 1, l’opportunitadi razionalizzare le modalita di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella promozione della Conferenza. – sull’emendamento 1.45 parere contrario,

sull’emendamento 2.17 (testo 2) parere non ostativo, a condizione che sia previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni per la definizione delle modalita di accesso al Fondo straordinario ivi previsto; sugli emendamenti 2.212 e 2.213 parere contrario, in quanto la disposizione interviene in modo diretto in materia di formazione professionale, che, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione, rientra nella competenza esclusiva delle Regioni. sull’emendamento 6.9 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista viola la competenza legislativa delle Regioni in materia di formazione professionale; sull’emendamento 7.68 parere non ostativo, a condizione che sia previsto un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in sede di adozione del decreto ministeriale volto a definire condizioni, modalitae importi dei buoni orari per alcune categorie di soggetti svantaggiati; sull’emendamento 11.214 parere non ostativo, a condizione che la disposizione sia riformulata con una norma di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione, in analogia a quanto gia disposto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2010, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42; – sui restanti emendamenti parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali: risulta confermata la disponibilitadelle risorse del Fondo di rotazione per le politiche europee, utilizzate a copertura delle misure di cui agli articoli 1, comma 12, per quanto attiene all’impatto sull’indebitamento netto e sul fabbisogno delle spese da sostenersi con le predette risorse, viene confermata la relativa neutralita, in quanto l’articolazione temporale della spesa prevista per i nuovi interventi ela medesima di quella stimata nei tendenziali per le misure definanziate; con riferimento all’articolo 2, comma 9, che estende il periodo di utilizzo del credito di imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, si fa presente che tale disposizione non incide sui limiti del finanziamento, risultando esclusivamente finalizzata a consentire ai beneficiari l’effettiva fruizione dell’agevolazione in questione; in relazione all’articolo 9, commi da 13 a 16, ove si eliminano i limiti di eta ai fini della costituzione delle societaa responsabilita limitata semplificate, si ritiene che tale tipologia societaria non sia idonea a sostituire in tutto e per tutto le SRL ordinarie e che, pertanto, i relativi effetti finanziari saranno poco significativi; per quanto attiene all’articolo 11, commi da 2 a 4, il ricorso all’anticipazione di tesoreria costituisce una mera possibilitache, in ogni caso, verrebbe regolarizzata in tempi molto brevi; in relazione all’articolo 11, commi da 18 a 20, ove si modificano le percentuali di acconto a titolo di pagamento dell’IRPEF, dell’IRES le stime del Governo sono state elaborate considerando anche l’eventualita che i contribuenti calcolino l’acconto non solo con il metodo storico, ma anche con quello previsionale; risulta suffragata l’effettiva disponibilita` delle risorse indicate dall’articolo 12 come copertura del provvedimento in esame; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che: l’utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche europee a copertura delle misure di cui agli articoli 1, comma 12, lettera a), e 3, commi 1 e 2, non pregiudichi interventi giaavviati, in rapporto ai quali le risorse non sono state ancora formalmente impegnate, ma di fatto erano ad essi destinate; – l’articolo 7, comma 5, lettera b), recante l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari dell’Assicurazione sociale per l’impiego non comporti effetti negativi per la finanza, pubblica, posto che, a fronte del beneficio economico per il datore di lavoro, non viene corrisposta la prestazione al lavoratore dipendente e, altresı, non viene riconosciuta la contribuzione figurativa, in presenza di contribuzione effettiva versata a seguito dell’assunzione; – in merito all’articolo 9, comma 12, le spese sostenute dagli enti locali per lo svolgimento di attivitasociali rappresentino effettivamente una voce di limitata incidenza nel complesso delle spese di personale; dall’articolo 10, commi 5 e 6, sui requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilita in favore dei mutilati e degli invalidi civili, non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una norma che conferma, per via legislativa, la prassi amministrativa giaadottata dall’INPS; – in relazione all’articolo 11, commi 7 e 8, concernente le agevolazioni per la ricostruzione post sismica in Emilia, il nuovo articolo 6-novies del decreto-legge n. 43 del 2013 risulti conforme alla normativa europea, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 47, comma 3, della legge n. 234 del 2012, che prevede la necessaria autorizzazione della Commissione europea; in merito all’articolo 11, commi da 13 a 16, l’utilizzo di quota parte dell’anticipazione di liquidita, concessa alla Regione Campania in base all’articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, per il finanziamento del piano di rientro dal disavanzo sanitario, non incida negativamente

l’utilizzo dıquota parte degli stanziamenti del Fondo di rotazione per le politiche europee, a copertura delle misure di cui agli articoli 1, comma 12, lettera a), e 3, commi 1 e 2, potrebbe comportare, in sede applicativa, il rischio di una dequaliflcazione della spesa, derivante dallo storno di risorse di parte capitale per il finanziamento di interventi di natura corrente; – con riferimento all’articolo 7, comma 5, recante l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), pur prendendo atto delle rassicurazioni del Governo sull’assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, si rileva come tale norma potrebbe agevolare anche i datori di lavoro che avrebbero, comunque, assunto i lavoratori in questione, i quali sarebbero decaduti dal relativo sussidio; per quanto concerne l’articolo 9, comma 3, si segnala il carattere potenzialmente oneroso di tale norma, laddove essa, senza prevedere un tetto di spesa, aggancia la durata massima complessiva dei periodi di apprendistato a quella individuata in sede di contrattazione collettiva; in relazione all’articolo 11, comma 12, si osserva che la facolta di aumento delle addizionali IRPEF alle Regioni a statuto speciale viene concessa, dal capoverso articolo 3-ter, a regime, a fronte di un pagamento dei debiti della pubblica amministrazione di carattere una tantum; si osserva, inoltre, sempre in relazione al medesimo articolo 11, comma 12, capoverso «Art. 3-ter», che l’aumento dell’addizionale IRPEF, concesso alle Regioni a statuto ordinario in ragione dell’applicazione dell’intera normativa riguardante il federalismo fiscale, non appare coerente in relazione alle Regioni a statuto speciale, alle quali non si applica integralmente tale disciplina, con particolare riferimento alla definizione dei costi e dei fabbisogni standard; per cio` che riguarda l’articolo 11, commi 22 e 23, che introduce l’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, si rileva come la Relazione tecnica non fornisca la fonte dei dati riportati, ne´ chiarisca in base a quali parametri, ovvero trend osservati, si sia giunti ad ipotizzare un mercato del settore di 200 milioni di euro a partire dal 2014. Inoltre, non sembra che si sia tenuto conto di possibili effetti disincentivanti, in relazione alle ricadute sul prezzo derivanti dall’imposta introdotta».

trasmessi dall’Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.22, 1.42, 1.5000/16, 1.5000/17, 1.5000/18, 1.5000/21, 1.5000/22, 1.5000/23, 1.5000/24, 1.5000/25, 1.5000/26,

2.3, 2.11, 2.19, 2.23, 3.6, 3.0.1, 3.0.2, 6.0.5, 6.9, 6.0.4, 6.0.6, 7.102, 7.79, 7.104, 7.105, 7.88, 7.95, 7.96, 7.111, 7.123, 8.0.1, 9.82, 9.0.1, 9.12, 9.34, 9.35, 9.66, 9.74, 10.9, 10.13, 10.17, 11.3, 11.4, 11.19, 11.21, 11.25, 11.53, 11.56, 11.58, 11.60, 11.7, 11.29, 11.35, 11.49 (ora 11.217), 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 1.200, 1.212, 1.214, 1.215,

2.208, 3.209, 3.212, 3.210, 3.0.200, 3.0.200 (testo 2), 5.200, 5.201, 6.0.200, 6.0.201, 6.0.202, 7.209, 7.211, 7.228, 7.229, 7.231, 7.232, 7.222, 7.223, 7.227, 7.230, 7.231, 7.219, 7.220, 7.224, 7.225, 7.226, 7.0.200, 9.201, 9.206, 9.202, 9.215, 9.220, 9.216, 9.218, 10.205, 10.206 e 10.0.200. Il parere edi semplice contrarieta sugli emendamenti 01.2, 1.43, 1.207, 2.8, 2.15, 3.1, 1.5000/28, 1.5000/29, 1.5000/34, 1.5000 (limitatamente alle parole «e sopprimere il secondo periodo» della lettera g)), 5.0.1, 6.10, 9.43, 9.57, 9.90, 9.94, 9.95, 11.20, 11.27, 11,46, 11.27, 11.37, 11.44, 11.48, 5.500/1, 11.0.501/1, 11.0.501/2, 11.0.501/3, 11.0.501 (testo corretto) (limitatamente al primo comma), 3.4 (testo 2), 1.226, 2.203, 2.204, 3.200, 3.201, 3.204, 3.206, 6.200, 6.201, 6.202, 6.204, 6.205, 7.206 e 9.214. In relazione all’emendamento 1.205 il parere di nulla osta econdizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: «nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16». Sugli emendamenti 1.217 e 1.220 il parere di nulla osta e condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, ad aggiungere le seguenti parole: «entro i limiti di cui al comma 4 del presente articolo e delle risorse di cui ai commi 12 e 16». Fino all’articolo 10 il parere edi nulla osta su tutti i restanti emendamenti. Il parere e sospeso sugli emendamenti 7.0.201 e 9.89. E[]altresı sospeso su tutti gli emendamenti, presentati solo all’Assemblea,

parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.202, 11.203, 11.204, 11.205, 11.217, 11.218, 11.224, 11.227, 11.229, 11.231, 11.233, 11.234, 11.235, 11.236, 11.237, 11.0.200, 11.200, 11.11, 11.201, 11.221, 11.222, 11.223, 11.228, 11.232 e 11.0.201. Il parere e` di nulla osta sui restanti emendamenti. Resta sospeso il parere sugli emendamenti 7.0.201, 9.8, 11.208, 11.210, 11.211, 11.225, 11.226, 11.219, 11.220 e 11.300, nonche´ sugli emendamenti presentati dal Governo». presentate dal Governo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall’Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.202,

A modifica del precedente parere, la Commissione esprime sulla proposta 11.25 parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: «50 milioni» con le seguenti: «10 milioni». E[]altresı revocato il precedente parere sull’emendamento 7.0.200, per il quale si esprime l’avviso di nulla osta. Il parere edi nulla osta sulle proposte 1.800, 1.801, 2.800, 3.800, 5.801, 9.800, 9.801 e 9.802. Rimane sospeso il parere sulle proposte 11.208, 11.210, 11.211, 11.225, 11.226, 11.219, 11.220, 11.300 e sui subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati dal Governo».

trasmessi dall’Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.800 (limitatamente alla lettera 11.210, 11.225, 11.226, 2.800/1, 2.800/2 e 7.800/1. Il parere di semplice contrarietae condizionato, ai sensi dell’articolo 81 medesima norma costituzionale, sulla proposta 9.802/1 alla soppressione, al capoverso: «188.» delle parole da: «ovvero» a: «studenti» e, altresı, alla soppressione del secondo capoverso: «Conseguentemente», recante la clausola di copertura. Il parere e di semplice contrarietasull’emendamento 11.219. Il parere e di nulla osta su tutti i restanti emendamenti». Onorevoli colleghi, la Presidenza, valutati gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge al nostro esame, riferiti agli articoli da 1 a 8, dichiara improponibili, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 6.204, 7.79, 7.217 e 7.218,

nell’emendamento, di operare una sorta di coordinamento tra i diversi interventi, quelli nazionali, ovviamente, ma anche quelli che si promuovono nell’ambito di ciascuna Regione. L’articolo 1, come e evidente nel testo, nel testo, mette in sinergia gli interventi dello Stato con quello delle Regioni, anche se, utilizzando le disposizioni che nello stesso articolo sono contenute, mette mette in sinergia le dotazioni finanziarie disponibili nell’ambito delle Regioni, cosıcome nell’ambito dello Stato. Quindi, si tratta di operare un coordinamento e, nell’ambito di questo coordinamento, rendere piu efficaci gli interventi che sono definiti dalle singole amministrazioni. In modo particolare, interessa anche la formulazione che noi diamo della platea dei destinatari, perche´ a nostro avviso una formulazione leggermente piutecnica piuttosto che

interveniamo solo su categorie svantaggiate, soprattutto su categorie dequalificate, rischiamo di avere una risposta negativa Siccome questo e un intervento di politica di sostegno all’occupazione che passa attraverso aiuti alle imprese, se noi obblighiamo all’assunzione di personale dequalificato, rischiamo l’inefficacia dell’intervento.

Presidente, con l’emendamento 1.200, e con altri, sempre riferiti all’articolo 1, si chiede di incentivare l’occupazione di lavoratori fino ai 35 anni attraverso interventi sul cuneo fiscale (tipo agevolazioni all’IRAP, all’IRPEF e contributive). Con questo emendamento, quindi, chiediamo un innalzamento dell’etafino ai 35 anni, perche´ questo decreto deve aiutare tutti i giovani, che noi consideriamo arrivare fino ai 35 anni, ma soprattutto a prescindere dal territorio di appartenenza. Vede, signor Sottosegretario, con questo decreto legge vengono discriminati, ma soprattutto umiliati, i giovani sopra i 30 anni. Una generazione che ha passato i 30 anni, con contratti a tempo indeterminato, viene umiliata due volte:

e volendo nel contempo invitare il Governo ad un ragionamento piucomplesso sul tema dell’occupazione giovanile over 30. Quindi, con un atto di responsabilita politica, voglio procedere al ritiro della mia proposta, ritenendo doveroso ragionare con il Governo su delle ipotesi di incentivo e di agevolazione all’occupazione, che si rivolgano anche ad un’altra fascia anagrafica non direttamente coinvolta in questo decreto. L’obiettivo, che spero venga condiviso anche dal Governo, equello di prevedere un piano urgente di intervento attraverso il quale modellare specifiche misure agevolanti per la fascia giovanile di eta maggiore con formazione universitaria, che, dati alla mano, risulta essere quella maggiormente colpita dalla crisi. Pertanto provvedo a depositare un ordine del giorno sulla questione, a firma mia e del collega Di Maggio.

illustro l’emendamento 1.211, che intende riconoscere un incentivo ai datori di lavoro nel caso di assunzione a tempo indeterminato

Presidente, senatrici e senatori, il provvedimento sul quale oggi ci apprestiamo a votare introduce delle misure che potremmo definire utili per il rilancio dell’occupazione giovanile, ma che al contempo presentano un grave difetto: sono caratterizzate da una sterilitadi idee. Cari colleghi, rielaborare per l’ennesima volta il contratto di apprendistato o introdurre norme per la stabilizzazione di qualche contratto precario non basta oggi per far ripartire l’Italia. Bisogna smettere di fare l’elemosina ai nostri cittadini e impegnarci per dare loro una prospettiva per il futuro. Ritengo con convinzione che sia preciso dovere della politica cominciare a risolvere alla radice il problema della crisi economica, partendo dal lavoro svolto in questo Parlamento e non invocando passivamente l’aiuto delle istituzioni europee. All’articolo 1 del decreto che oggi andiamo a convertire in legge vengono inseriti degli incentivi alla stabilizzazione dei contratti per i giovani tra i 18 e i 29 anni, cercando di convincere le aziende a rendere stabile il lavoro, anche in una situazione di instabilita diffusa del mercato. La nostra economia ha bisogno di ben altro per rialzarsi; una volta rilanciati i consumi e le esportazioni, le nostre aziende non avranno bisogno di incentivi per assumere nuovi giovani. E[]per questo che chiedo al Senato di approvare l’emendamento 1.213, da me presentato, che vuole rappresentare un piccolo punto di partenza per rilanciare il lavoro dei nostri giovani e al contempo promuovere il made in Italy nel mondo: un concreto impegno per far usufruire dell’incentivo previsto dall’articolo 1 anche quelle aziende che vogliono allargare il proprio mercato all’estero, andando a promuovere i nostri prodotti migliori made in Italy, che vantano una fama internazionale senza pari nei Paesi emergenti, che stanno dimostrando di apprezzare tantissimo la qualita artigianale e industriale italiana. Nell’emendamento eprevisto anche che sia il Ministero dello sviluppo economico ad individuare, mediante decreto, le modalita con cui le aziende potranno accedere all’incentivo. Potra, ad esempio, prevedere dei pacchetti standard suddivisi in categorie di prodotti a cui le aziende potranno fare riferimento per presentare il loro piano di promozione. Tale impostazione organica di esportazione del prodotto italiano potrebbe potrebbe permettere di promuovere anche delle offerte low cost, aumentando esponenzialmente la domanda e quindi la produzione, rigorosamente italiana. I nostri giovani potranno presentare i prodotti made in Italy in fiere ed expo valorizzando il patrimonio artistico e paesaggistico collegato al turismo culturale, le specialita gastronomiche e alimentari richieste in tutto il mondo, la grande tradizione italiana legata alla moda e all’industria calzaturiera. Prevedendo un incentivo di questo tipo non facciamo solo un favore alle aziende italiane e ai giovani, ma facciamo qualcosa di nuovo per l’Italia. Potremo cominciare a seminare per poi raccogliere in futuro, una cosa che in questi ultimi anni non siamo riusciti a fare. (Applausi della

1.42, 1.43 e 1.44 sono preclusi perche´ sul tema e stato presentato dal Governo l’emendamento 1.801 che riscrive la procedura per l’accesso agli incentivi e tutti questi emendamenti fanno riferimento a modifiche di regole della procedura.

ritiro l’emendamento 1.201

Cosı` oltre agli scripta rimangono anche gli audita. quindi la riformulazione del testo consiste nell’avere il testo depennato cosıa penna, rigo piu

l’emendamento 1.800 riscrive la lettera c). PRESIDENTE. Va bene. E[]un chiarimento che forse puo aiutarci nell’andare avanti.

per i quali eprevisto che il datore di lavoro versi almeno 156 contributi giornalieri in un anno solare, a quelli a tempo indeterminato. Infatti, in agricoltura

dobbiamo andare a farlo tutti insieme. Andiamo a spiegare come mai ancora non riusciamo a votare certi provvedimenti per i cittadini e invece ci blocchiamo su un articolo,

E poi soprattutto la invito, eventualmente, a fare una lezione tecnica sulla votazione, perche´ continuano a sbagliarsi a votare. Credo che questo meriti la nostra considerazione: se non sono buoni neanche a votare, non so cosa ci vengano a dire.

E[]un tema a cui il mio Gruppo tiene molto. Si tratta della possibilita di considerare misure diversificate, in questo caso tra i generi, con riferimento

mettano in evidenza con assoluta chiarezza un differenziale di genere importantissimo. Noi avevamo predisposto un emendamento, che certamente aveva bisogno di ulteriori approfondimenti perche´ l’attuazione di meccanismi di discriminazione positiva negli incentivi e oggettivamente di difficile formulazione. Per questo motivo ritiriamo il nostro emendamento, ma chiediamo al Governo di impegnarsi a valutare, ogni qualvolta dispone misure di politica del lavoro e, soprattutto, misure relative all’occupabilita`, il fatto che gli effetti delle misure non sono identici sui due generi, perche´ diverse sono le condizioni di partenza nel mercato del lavoro degli uomini e delle donne.

E[]vero che i nostri giovani del Nord sono pronti ad emigrare, a lasciare il proprio territorio e la propria famiglia pur di cercare un lavoro, contrariamente ai giovani disoccupati del Mezzogiorno che preferiscono restare disoccupati, inoccupati ed assistiti piuttosto che lasciare la terra d’origine.

Senatrice Bellot,

si stanno sovente violando articoli del Regolamento, e – cioche mi preoccupa – la prassi parlamentare, perche´ quando si adotta una regola, seppure nuova, essa

la norma e molto chiara nel precisare che l’intervento deve essere limitato a dichiarare il voto favorevole, contrario

Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il nostro ordinamento prevede, in numerosissimi casi, la possibilitache sia il contratto collettivo a temperare le asperita di norme che vengono, in un certo senso, tagliate a colpi d’accetta a livello nazionale ma che possono, in certe circostanze, rivelarsi troppo rigide.

relative all’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato, nelle quali la ragione della restrizione posta dalla norma statuale viene meno nella situazione concreta. La funzione di adattamento eaffidata alla contrattazione collettiva nazionale. Chiediamo che si valuti con attenzione la possibilita di questa forma di flessibilizzazione.

l’ordine del giorno G2.100, proposto dal senatore Russo, il Governo esprime favorevole con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare la possibilita`, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in armonia con la disciplina generale in tema di assunzioni».

su quale base del nostro Regolamento, regolarmente, possiamo correggere il nostro voto o segnalare che non abbiamo votato? (Applausi dai Gruppi nell’ultimo voto di fiducia giustamente – ripeto giustamente – lei non mi ha fatto votare perche´ sono entrato in ritardo in Aula, anche se non ero in spiaggia ma in sala Zuccari ad un convegno. Giustamente, ripeto, non mi ha fatto votare. Per quale motivo e su quale base del Regolamento qui ogni volta si cambia il voto o si dice di non aver potuto partecipare, soprattutto quando questi voti sono nominali e registrati?

Viene dichiarato il voto e resta agli atti. Senatore, lei sa che il risultato non viene modificato: resta agli atti il voto, ma il risultato e` quello elettronico. Quindi non influenza…

ho detto che lo doveva fare suo prima che fosse ritirato. Presidente, mi scusi, se il collega Zeller avesse mantenuto l’emendamento, io avrei aggiunto la firma.

le dico che non mi piaceva essere preso in giro, da questa gente qui, e non e` giusto che dentro quest’Aula queste persone ci prendano in giro.

sulla procedura web messa a disposizione dal Ministero. In questo caso, quello che chiediamo e`: volete voi amministrazioni, in questo periodo, prendere persone a fare i tirocini? Bene, perfetto: ma mettiamoli esclusivamente in quegli uffici ad aiutare le pubbliche amministrazioni a caricare i dati e a pagare le nostre imprese. Questo stiamo chiedendo con questo emendamento. (Applausi

La filosofia che edentro questo articolo e agli emendamenti che sono stati proposti va esattamente nel senso contrario: una legalizzazione dello sfruttamento del lavoro giovanile, esattamente il contrario di quello che noi dobbiamo chiedere. Ecco perche´ io voterocontro questo emendamento e votero contro tutti gli emendamenti che hanno questo tipo di ispirazione.